Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, nonché in analogia al parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Circoscrizione estero-ripartizione Europa, a seguito delle dimissioni del senatore Nicola Paolo Di Girolamo, che l'Assemblea ha accolto nella seduta antimeridiana odierna, ha riscontrato, nella seduta del 3 marzo 2010, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali all'interno della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Raffaele Fantetti. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore Raffaele Fantetti. Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro",

*relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, illustri colleghi, giunge alfine in quarta lettura al Senato il collegato lavoro alla finanziaria. La Camera dei deputati ha operato interventi mirati e selettivi sul testo così come da noi licenziato, i principali dei quali sono due. Il primo intervento riguarda la materia della conciliazione e dell'arbitrato, regolato dall'attuale articolo 31 della disposizione che stiamo esaminando. La modifica apportata dalla Camera, che intercetta sollecitazioni fatte fatte proprie dai colleghi e dagli amici dell'opposizione, cambia il regime di entrata in vigore in termini di concreta operatività della norma. Infatti, laddove era prevista una finestra di 18 mesi, al termine della quale sarebbe divenuta automaticamente effettiva l'apparecchiatura normativa predisposta dal testo, oggi è invece previsto che, dopo 12 mesi, il Ministero del lavoro senta le parti sociali e, sulla base degli esiti della consultazione realizzata con le medesime parti sociali, disponga autonomamente le modalità di implementazione del collegio di conciliazione e dei collegi arbitrali, così come rinnovatamente disegnati dalla norma. L'altra modifica apportata dalla Camera al nostro testo riguarda la materia dell'apprendistato. È inutile celare che questo tema ha suscitato qualche polemica. Si tratta di una disposizione la quale interviene con un'attitudine specificativa rispetto ad una delle tre forme di apprendistato introdotte nella nostra legislazione dalla legge Biagi. In particolare, si fa riferimento a quel tipo di apprendistato funzionale all'espletamento della missione di istruzione e di formazione (in qualche modo, è la forma di apprendistato nella quale l'equilibrio tra la causa di lavoro e quella di formazione, tipica di un contratto che tutta la dogmatica riconosce appartenere alla categoria dei contratti a causa mista, vede una sorta di concentrazione della trazione Il ruolo di questo istituto è quello di accompagnare i ragazzi al completamento del percorso dell'obbligo scolastico, sul quale era intervenuta la legislazione del Governo Prodi stabilendo un nuovo limite di età, che non viene toccato dalla norma così come novellata dalla Camera. La norma novellata dalla Camera, infatti, si limita a intercettare quei casi nei quali, essendosi verificato un fenomeno di diserzione dall'obbligo scolastico, al giovane sia consentito di anticipare di un anno (e quindi al compimento del quindicesimo anno di età) l'accesso a a quella particolare tipologia di apprendistato che è l'apprendistato funzionale all'espletamento dell'obbligo di istruzione. Quindi, in qualche misura si tratta di intercettare l'area grigia e opaca, spesso contaminatamente preda del lavoro nero o, peggio, del lavoro criminale, che al Sud, ma anche al Nord, è significativamente espressiva di un disagio sociale e di *dropout*, che vanno invece restituiti a un accesso regolare e trasparente al mercato del lavoro. Se questi sono i due interventi principali disposti dalla Camera, altri ve ne sono che hanno marginalmente rimodellato l'impianto e che, quindi, mi limito a ricordare ai colleghi. L'articolo 1 è intervenuto sulla delega sui lavori usuranti, introducendo un criterio di priorità tale per cui, a parità di risorse disponibili, prevalga prima l'ordine di maturazione dei requisiti e poi di decorrenza delle domande. Nell'articolo 2 è stato introdotto, a seguito dello *splitting* istituzionale tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, un recepimento di questa avvenuta distinzione

All'articolo 21, che regolava la materia dei comitati di tutela e promozione delle pari opportunità nel lavoro pubblico, è stata molto opportunamente inserita la doverosità della collaborazione di questi comitati con la Consigliera nazionale di parità ed è stato stabilito, come norma di prudenza finanziaria, il fatto che tutti gli interventi di rimodellamento organizzativo debbano essere implementati senza oneri. inoltre soppresso l'articolo 25, relativo ai certificati di malattia. Per quel che concerne l'articolo 32, relativo alle clausole di decadenza, sono state introdotte, con funzione specificativa, due ipotesi, l'una relativa ai casi di cessione del contratto di lavoro (*ex* articolo 2112 del codice civile), l'altro relativo agli accertamenti del reale titolare del contratto di lavoro medesimo. Agli articoli 42 è 43, relativi, rispettivamente, alle comunicazioni dell'impresa di assicurazione all'INPS e all'iscrizione o cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali, è stata introdotta ancora una volta una clausola di guarentigia finanziaria prevedendo la doverosa non onerosità degli interventi. Sull'articolo 46 si è intervenuti rimodulando la durata delle deleghe: è stata cioè introdotta una norma per la quale, per tutte le deleghe previste dall'articolo - quindi, quella relativa agli ammortizzatori sociali, al lavoro femminile, all'apprendistato, ai servizi per l'impiego, agli incentivi per l'occupazione

All'articolo 48 sono state disposte modifiche rispetto alla *machinery* delineata dal Senato, lungo queste traiettorie: il rafforzamento della borsa lavoro; la semplificazione della procedura di operatività delle agenzie di somministrazione; il rafforzamento del ruolo di garanzia svolto dal contratto collettivo nazionale di lavoro nella definizione del quadro di operatività per i fondi bilaterali. Infine, è stata soppressa la deroga per via contrattuale alle norme sull'apprendistato, questa norma essendo stata recepita in finanziaria. Presidente)*. Concludendo, credo si possa esprimere un giudizio positivo su questo collegato lavoro, che, coerentemente e conformemente al fatto di essere un collegato alla finanziaria, reca una normativa plurale plurale che, nell'approccio alla grande crisi e all'impatto che la stessa ha sugli scenari sociali, occupazionali ed economici del nostro paese, segnala un approccio molto pragmatico, pragmatico, segnala che la contiguità al punto del fare è l'area elettiva per gli interventi di correzione degli andamenti economici. È in qualche modo un provvedimento che consapevolmente, programmaticamente, deliberatamente assume un approccio rapsodico, nel senso che coglie tutte le opportunità di modulazione degli interventi senza restare necessariamente prigioniero del loro astratto *frame* generalista. Questa è una delle condizioni che hanno garantito il successo complessivo delle politiche... *(Brusìo. Richiami del Presidente)* ... del nostro Governo rispetto alle manifestazioni della grande crisi e che oggi consente di coagulare e condensare una piattaforma per la ripresa. L'ultimo tratto dal punto di vista metodologico è quello della progressività, quello che, scherzosamente con il collega Ichino, in altra circostanza, avevamo definito l'approccio della stratificazione virtuosa. Questo è un provvedimento che speso ha visto suoi pezzi asportati e collocati in altri provvedimenti, proprio perché la necessità di un approccio assolutamente modulato e flessibile... *(Brusìo)*. PRESIDENTE. Volete far parlare tranquillamente il collega? Devo chiamare ora uno per uno, senatrici e senatori che non consentono al relatore di svolgere la relazione? *relatore*. Ringrazio il signor Presidente per l'intervento di supporto che colgo, in qualche misura, anche come una sollecitazione a concludere. Abbiamo fatto un cenno rapidissimo al dato metodologico. Sul tema dei contenuti credo si possa dire

sui presupposti tecnici assunti nelle decisioni delle parti contrattuali - diventa un *driver* di coesione sociale, così come sull'altro versante la coesione sociale è il frutto degli interventi di valorizzazione dell'autonomia delle parti sociali (si pensi solo alla conciliazione e all'arbitrato). È evidente che, in un momento di crisi come, questo affiancare, giustapporre alla via giudiziaria

vettore di qualità competitiva per il nostro sistema economico e sociale. Credo che ora sia il collega Saltamartini a completare l'illustrazione per quanto concerne la parte relativa al lavoro pubblico.*(Applausi

semplicemente apportato alcuni aggiustamenti di carattere prevalentemente letterario e semantico. Vorrei però, Presidente, ricordare qui che anche in questo testo continua ad apparire questo errore sul nove latino, che continua ad essere riportato come 9-*nonies* essere invece che 9-*novies*. L'avevo già fatto presente in 1a Commissione: questo errore nasce da una circolare allegata alla legge n. 400 del 1988 dell'allora sottosegretario Amato e sostanzialmente

Detto questo, la norma che riguarda la 1a Commissione affari costituzionali e in particolare la parte relativa al regime del pubblico impiego è una previsione che concerne il conferimento di una delega legislativa al Governo per la ristrutturazione del sistema previdenziale ed assistenziale del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

colleghi, vi chiedo un momento di attenzione perché la questione pregiudiziale che rapidamente illustrerò è di rilevantissima gravità. nasce probabilmente da un equivoco in cui è caduta la Camera nell'introdurre nel testo della legge, tra le norme che si applicano anche in materia di controversie di pubblico impiego, l'articolo 412 del codice di procedura civile. Probabilmente chi ha inserito l'articolo 412 pensava ancora al vecchio articolo 412, che tratta di conciliazione; i lavori della Camera sembrano proprio indicare questo. E lo stesso Presidente della Commissione lavoro del Senato

cambia la numerazione e adesso al 412 sta l'articolo che regola l'arbitrato. Quindi, se la norma venisse approvata così com'è,

le controversie - leggo testualmente dall'articolo 63 del testo unico richiamato - che riguardino l'assunzione al lavoro, il conferimento e revoca di incarichi dirigenziali, la responsabilità dirigenziale, l'indennità di fine rapporto, anche quando vengano in questione atti amministrativi presupposti. In questo caso - dice l'articolo 63 del disapplica l'atto amministrativo. Quindi, l'arbitro potrà disapplicare l'atto amministrativo. Questo contrasta in modo plateale innanzitutto con l'articolo 97 della Costituzione che stabilisce, tra gli altri, il principio dell'accesso agli uffici pubblici per concorso. Qui l'arbitrato consentirà di eludere ed aggirare la norma sul concorso; ma consentirà l'arbitrato anche su altre cose che sono vistosamente non suscettibili di essere devolute a un arbitro.

meriterebbe davvero un ulteriore brevissimo passaggio alla Camera dei deputati, anche solo per correggere questo strafalcione - ripeto - involontario, perché se guardate i lavori della Camera sembra proprio che anche i deputati siano caduti in questo equivoco.

finestra"). Ricordo che sulla questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, si svolge un'unica discussione, durante la quale può intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Chiedo ai colleghi, soprattutto al Governo e alla maggioranza, di prestare qualche minuto di attenzione sul tema che il professor Ichino ha appena sollevato in Aula.

vorrei leggere all'Aula il testo del parere della Commissione bilancio, approvato dalla maggioranza della Commissione bilancio stessa con il nostro voto contrario, perché abbiamo chiesto di esprimere parere contrario sull'articolo 31, La maggioranza non ha accolto tale proposta, signor Presidente, ma se lei esamina il testo del parere della Commissione bilancio troverà questa frase: «parere non ostativo sul testo, osservando che dalla modifica contenuta nell'articolo 31, volta a recepire nella pubblica amministrazione la risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro, potrebbero determinarsi effetti finanziari negativi».

riconosciuto come la questione da noi posta, cioè di possibili effetti finanziari negativi sul bilancio determinati da questa innovazione legislativa, sia assolutamente fondata. Vorrei, non avendo la stessa precisione e la stessa padronanza delle tecnicalità che ha il professor Ichino sull'argomento, andare all'essenziale. Signor Presidente, di cosa si tratta? In buona sostanza, l'innovazione introdotta dalla Camera consente di utilizzare soluzioni arbitrali delle controversie di lavoro nella pubblica amministrazione. amministrazione. Non ricorrerò alla cronaca di questi giorni per sostenere la tesi che nella pubblica amministrazione italiana e soprattutto nel comportamento di certa componente della sua dirigenza sono presenti - chiamiamole così - vistose anomalie, fonte di particolari preoccupazioni. Ma vorrei andare all'essenziale. Se questa norma rimane così com'è, cosa può accadere? Ad esempio, io sono un dipendente pubblico ho intenzione di tentare la scalata ad un ruolo dirigente nell'amministrazione nella quale lavoro: che cosa faccio? Promuovo una controversia. So benissimo che è completamente infondata, so benissimo, in buona sostanza, che non ho alcuna possibilità di risultare prevalente nella controversia che sto promuovendo, ma ho un grande vantaggio: sono amico del dirigente della pubblica amministrazione dell'ufficio nel quale lavoro. Cosa può a quel punto accadere, signor Presidente (e non sto esagerando, sto descrivendo quello che secondo me può accadere e accadrà se lasciamo la norma così com'è)?

Ora, è del tutto evidente che se mi metto d'accordo, visto che sono amico, con il dirigente della pubblica amministrazione possiamo far nominare un collegio arbitrale che in partenza dà ragione al sottoscritto, anche se la "ragione" non la ho. Risultato: chi paga?

La finanza pubblica italiana è esposta da questa norma ad un rischio veramente molto serio.

una norma di cui la maggioranza della Commissione bilancio, pur orientata, per ragioni procedurali - cioè non tornare alla Camera - a non dare un parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione, ha tuttavia dovuto scrivere nel parere

per risolvere controversie che riguardano l'assunzione nel posto di lavoro. Già abbiamo una pubblica amministrazione alla quale non si accede più per concorso;

Guardate che si tratta di una norma potenzialmente devastante dell'intero impianto della finanza pubblica italiana, dal lato, ancora una volta, dell'aumento della spesa corrente primaria. È qualcosa che merita attenzione, colleghi, al di là della pregiudiziale di costituzionalità. Discutiamo una volta senza il velo del preconcetto: sapete che abbiamo ragione, che l'argomento portato dal professor Ichino è

che dovrebbero preoccupare, in primo luogo, chi sta esercitando l'azione di governo e intende esercitarla fino al 2013 con risultati positivi. Ma dove va a finire la riforma della pubblica amministrazione, che io chiamo legge Brunetta-Ichino, se si applica questo principio? Vi rendete conto di quali sono i possibili effetti di annichilimento di quella innovazione, che pure è di grande portata? Vi prego, al di là di maggioranza e opposizione, di tener conto di questi argomenti e di accettare di modificare il testo sul punto che riguarda l'espunzione da questa legge del riferimento all'articolo 412 del codice di procedura civile.

liberista impone, come ritmo fondamentale, alla società una direzione, che è quella di utilizzare le risorse pubbliche per farle finire in tasche private.

In nome del liberismo, in nome dell'arbitrato e in nome della maggiore libertà economica voi spostate d'un colpo i rapporti di forza interni al mercato del lavoro con una virulenza inaccettabile;

furioso liberismo che intriderebbe questa norma facendo presente che la clausola arbitrale è prevista negli accordi confederali dei contratti collettivi ed è uno strumento agevole per risolvere in tempi brevi e accettabili controversie che, se seguissero la strada giurisdizionale prenderebbero un tempo sicuramente maggiore. Tornando alle osservazioni di ordine tecnico svolte dal senatore Ichino e dal senatore Morando, voglio far presente che nel

Ci lamentiamo sempre che i due settori costituiscono una sorta di sistema duale, spesso confliggente e che spesso non produce quella normale armonia che ci dovrebbe essere.

in essa previsto che la giurisdizione, in alcuni casi, possa essere affidata ai cosiddetti privati. Perché non allargare questo strumento, che per controversie di genere diverso è tuttora vigente, anche al settore pubblico? che le argomentazioni dei senatori Ichino e Morando in ordine alle conseguenze che potrebbero derivare da questo sistema non siano assolutamente fondate e mi chiedo, in particolare, perché temere che questo possa comportare un onere maggiore e non fare, invece, lo stesso ragionamento nel caso in cui permanesse la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare è, nella sostanza, quello approvato in questa stessa Aula pochi mesi fa, e questo, ovviamente, non porta certo a considerazioni positive. Le modifiche apportate al provvedimento da parte della Camera dei deputati sono state, di fatto, poche. Di esse quasi nessuna è sostanziale, mentre quasi tutte sono peggiorative di un testo già di per sé pasticciato, risultato di quel vero e proprio assalto con il quale la maggioranza, nel corso della precedente lettura al Senato, inserì un'accozzaglia di norme sugli argomenti più disparati trasformando il provvedimento in discussione in un mostro di oltre cinquanta articoli, privo di qualunque coerenza e sistematicità. Il principale rilievo critico, a proposito delle modifiche apportate alla Camera, riguarda la norma sull'apprendistato di cui al comma 8 dell'articolo 48. Il contenuto della norma è noto: si prevede che il contratto di apprendistato possa assolvere all'obbligo scolastico. La specifica disposizione così recita: «l'obbligo di istruzione (...) si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003». Di fatto, si abbassa in modo surrettizio il limite scolastico obbligatorio, attualmente di sedici anni, consentendo, a chi lo volesse, di iniziare a lavorare come apprendista già a quindici una pessima norma per almeno tre ordini di motivi che cercherò brevemente di illustrare. Anzitutto, si tratta di una norma anacronistica. Va ricordato infatti che il prolungamento a dieci anni del periodo di istruzione obbligatoria (e il conseguente elevamento a 16 anni dell'età per l'accesso al lavoro) è stato introdotto in Italia soltanto a fine 2006 dal Governo Prodi. Tuttavia, se allarghiamo lo sguardo all'Europa, rileviamo che purtroppo, anche in questo caso, il nostro Paese è stato tra gli ultimi ad adottare una simile normativa, mentre in gran parte degli altri Paesi l'obbligo scolastico fino a 16 anni era già previsto da molto tempo. Inoltre, a tutt'oggi l'orientamento maggioritario, sempre all'interno dell'Unione europea, è di elevare ulteriormente il limite dell'obbligo scolastico portandolo a 18 anni. Il provvedimento in esame, invece, si muove esattamente nella direzione opposta. secondo luogo, si tratta di una norma disorganica e irrazionale. Disorganica perché, appena due articoli prima (precisamente all'articolo 46, comma 1, si prevede una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati al riordino, tra l'altro, proprio della normativa in materia di apprendistato. Irrazionale perché, esattamente come nel caso della reintroduzione del famigerato *staff leasing* (i cosiddetti contratti di lavoro in affitto), non si comprende la necessità di una simile norma se non per motivi puramente ideologici. Infine, e veniamo al terzo (e più grave) motivo, è una norma potenzialmente assai dannosa per il futuro dei nostri giovani. Secondo quanto dichiarato più volte dai rappresentanti del Governo, lo scopo dell'introduzione all'articolo 48 del nuovo comma 8 non consisterebbe nell'anticipare l'età del lavoro, ma sarebbe volta a recuperare tutti coloro che non proseguono gli studi, inserendoli in una nuova modalità di apprendimento direttamente calata nel contesto lavorativo. L'Italia registra in effetti un indice di abbandono dell'istruzione scolastica pari a circa il 22 per cento, tra i più elevati d'Europa. Esso costituisce un ulteriore handicap nel conseguimento degli obiettivi previsti dal Trattato di Lisbona: la riduzione e la prevenzione della dispersione scolastica, l'incremento del numero dei laureati e diplomati, l'elevazione della qualità dell'istruzione e della formazione e l'ampliamento dell'obbligo scolastico e formativo. Un problema grave e concreto, dunque, quello dell'abbandono scolastico, che colpisce soprattutto il settore dell'istruzione tecnica e professionale. Ora quale sarebbe la risposta a questo problema? Un ulteriore abbassamento dell'età scolastica? È ovvio che il risultato di tutto ciò rischia di essere l'esatto opposto dell'obiettivo dichiarato: si rischia cioè un drastico innalzamento del livello di abbandono scolastico. Anzitutto i fattori di rischio che favoriscono l'abbandono scolastico sono riconducibili sicuramente a fattori socio-ambientali ed anche personali e familiari. Consegnare i giovani di 15 anni ai sistemi formativi extrascolastici significa lasciarli da soli e con tutte le problematiche che si trascinano dietro. Non è di certo il mondo produttivo a dover risolvere il problema dell'abbandono scolastico: è la scuola, che se ne è fatta sempre carico, e deve continuare ad essere la scuola a mettere in atto tutte le strategie possibili per fare in modo che i ragazzi non abbandonino la scuola stessa. dunque ripensare al sistema dell'istruzione e della formazione e al rapporto che questo deve avere con il mondo del lavoro. Bisogna aumentare l'offerta formativa, perfezionare le scuole professionali e il triennio degli istituti tecnici. Se non sarà affrontato il nodo della formazione, che non può essere lasciato alle aziende, a cui mancano anche le strutture per realizzarla, assisteremo ad un ovvio impoverimento non solo culturale dei nostri ragazzi, ma anche (ed è questo, forse, il punto più grave) professionale. Avremo semplicemente un esercito di manodopera generica in un mercato del lavoro che invece chiede sempre di più manodopera specializzata. In Italia l'apprendistato, come modalità di accesso al lavoro, ha incontrato grandi difficoltà proprio nell'attuazione della frequenza alle ore di formazione. E, ancora una volta, di questa tipologia di contratto traggono beneficio quasi esclusivamente le aziende, che risparmiano sia sul salario erogato, visto che gli apprendisti sono inquadrati ad un livello inferiore rispetto agli altri lavoratori e ricevono comunque una minore retribuzione anche quando l'inquadramento è lo stesso, sia dal punto di vista previdenziale, poiché è lo Stato a pagare i contributi obbligatori. Non è un caso, insomma, che, nel corso delle audizioni in Commissione, siano state espresse critiche pressoché unanimi a quanto previsto dall'articolo 48. Per quanto ci riguarda, come Gruppo Italia dei Valori, la nostra posizione in merito è netta e senza mezzi termini: il comma 8 dell'articolo 48 va semplicemente soppresso. Per concludere, svolgo alcuni brevi accenni su due ulteriori punti di criticità di questo provvedimento: le deleghe al Governo in materia di ammortizzatori sociali (articolo 46) e di lavori usuranti (articolo 1), e la cosiddetta norma interpretativa di cui all'articolo 20. Quanto all'articolo 1, sono assai forti le perplessità in merito ai meccanismi di priorità nella liquidazione dei trattamenti pensionistici. Il meccanismo previsto, infatti, potrebbe comportare che anche chi abbia maturato i requisiti agevolati potrebbe non vedersi riconosciuto il trattamento pensionistico perché, per una mera questione di termine di presentazione della domanda, potrebbe trovare le risorse esaurite. Per quanto riguarda invece le deleghe al Governo per il riordino della normativa in tema di ammortizzatori sociali - come del resto era già stato sottolineato nel corso del precedente esame al Senato l'attuale situazione di crisi economica e le conseguenze che essa ha avuto sull'occupazione rende non ulteriormente rinviabile quanto pattuito con il Protocollo sul welfare.

un breve accenno sull'articolo 20, che verrà poi illustrato in modo migliore dal collega Pardi. Si tratta dell'ennesima norma volta a bloccare la giustizia che, nel caso specifico, è quella militare. Questa finta norma interpretativa, sulla cui introduzione dovremmo fare tutti ammenda, regala l'impunità a coloro che avrebbero dovuto vigilare sulla salute dei propri uomini. In conclusione, Presidente, mi si lasci fare una considerazione sull'articolo 31 in materia di arbitrato e conciliazione. Come avevamo già avuto modo di sottolineare durante il precedente passaggio, questa norma, introducendo un vero e proprio arbitrato obbligatorio risulta essere gravemente lesiva dei diritti dei lavoratori e costituisce di fatto un aggiramento dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. cioè, cercando di realizzare in modo indiretto quell'operazione di stravolgimento del diritto dei lavoratori che non vi era riuscita nel 2002. Proprio per questo vi chiediamo di ritirare il provvedimento visto che questa norma vergognosa non è più modificabile. *(Applausi

Signor Presidente, voglio attirare l'attenzione su un argomento che in questo provvedimento

gerarchie militari di alto livello, che di fatto vengono scagionate, sollevate dal peso del rinvio a giudizio da parte del tribunale di Padova riguardo

primo luogo, ci si è già chiesti più volte perché mai argomenti di questo tipo debbano essere infilati di soppiatto in provvedimenti che in realtà si occupano di tutt'altro. È un'abitudine alla quale non ci abitueremo mai

gerarchie militari dell'Esercito a proposito dell'uranio impoverito. I due elementi - amianto, da una parte, e uranio impoverito, dall'altra - costituiscono una prova sgradevole e irrimediabile dell'atteggiamento del tutto parziale che la maggioranza e il Governo hanno nei confronti di questi temi così terribili. In sintesi, i soldati italiani vengono imbarcati in navi con l'amianto; vengono inviati in missioni all'estero dove vengono contaminati dall'uranio impoverito la loro vita professionale di militari viene incrinata o troncata per via dei danni irrimediabili alla salute. tutto quello che il Governo e la maggioranza sanno fare è quello di proteggere le alte gerarchie militari che non hanno svolto con oculatezza i compiti di protezione nei confronti dei loro soldati.

è vero, perché se la Patria invia in condizioni difficili i propri militari una parte di cura la deve affrontare, e su questo la Patria è estremamente colpevole perché non ha mai preso le misure dovute. Ricordo infatti che c'è un'inadempienza sostanziale, al di là dei cavilli di legge, che va tutto a danno dei militari delle basse gerarchie mentre solleva dal loro peso soltanto le alte gerarchie. Si ravvisa una lesione dell'uguaglianza e anche un atteggiamento incline a pensare che, tutto sommato, chi decide, per condizioni di vita difficili e di scarso reddito, di condurre quel tipo di vita, in realtà è meglio se ci ripensa e non si espone a quel tipo di rischi.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo colleghi senatori, il provvedimento in esame contiene importanti innovazioni per il mondo del lavoro privato e pubblico. Il Senato in prima lettura aveva apportato rilevanti modifiche; ricordo brevemente la questione della rappresentatività sindacale. La Lega è riuscita a far riconoscere il principio che un sindacato, per essere tale, deve essere realisticamente rappresentativo dei lavoratori, dei loro interessi, delle loro istanze, dei loro diritti, e deve essere radicato nel territorio e non - sicuramente - nei palazzi romani. Inoltre, l'inserimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle disposizioni di cui all'articolo 19 del provvedimento, in materia di specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere, dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale,

sull'articolo 2 per recepire l'avvenuta separazione del Ministero della salute da quello del lavoro; a quelle, sempre sull'articolo 2, volte a sottolineare

a garantire che le misure che devono introdurre le pubbliche amministrazioni non debbano comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La modifica che riteniamo più importante, comunque, è l'introduzione di una delega al Governo per l'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale dei Vigili del fuoco, finalizzata ad equiparare il trattamento di infortunio invalidante e grave malattia tra Vigili del fuoco volontari e in servizio permanente, nonché il trattamento pensionistico per i familiari dei volontari deceduti per cause di servizio a quello del personale permanente. Ringrazio i colleghi dell'altro ramo del Parlamento per questa modifica ricordo che questa rappresenta una battaglia storica della Lega, portata avanti per un criterio di giustizia ed equità. Dinanzi ad eventi tragici come un decesso ed un infortunio, le persone che volontariamente si mettono a disposizione della collettività non possono essere trattate differentemente dal personale permanente, perché hanno pari dignità e pari diritti. Infine, voglio soffermarmi sulla modifica di cui all'articolo 48 che prevede che l'ultimo anno dell'obbligo formativo possa essere soddisfatto

e l'abbandono scolastico, bensì il contrario: parliamo di una misura volta a realizzare un ponte formativo con il mondo del lavoro, un'opportunità in più per il giovane studente, che potrà scegliere se proseguire il tradizionale percorso di istruzione scolastica oppure avvicinarsi, già all'età di 15 anni, al mercato del lavoro ed alla realtà aziendale. Ricordando, altresì, l'importanza che ricopre l'articolo 1 del provvedimento, attesa da anni dai lavoratori che hanno svolto mansioni usuranti, spero

esempio della cattiva qualità normativa e legislativa di questa nostra legislatura, perché assembla in maniera incoerente una serie di questioni che nulla hanno a che vedere con il titolo e le finalità originarie della legge. La seconda questione riguarda l'insufficiente precisazione della definizione dei criteri di accesso alla quiescenza anticipata per i lavoratori impegnati nei lavori usuranti

importante è quello dell'ulteriore estensione degli ambiti di applicazione dell'arbitrato per equità alle controversie di lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione, oltre all'ulteriore proroga dei termini di 24 mesi dell'esercizio della delega nel frattempo scaduta su temi importantissimi, quali la riforma degli ammortizzatori sociali, le politiche attive per l'accesso al mercato del lavoro, l'occupazione femminile e le pari opportunità, che dimostra, a nostro avviso, l'intenzione del Governo di svuotare il contenuto originario di questa delega e di non attuarla nella sostanza. Il punto su cui però

assolutamente imprecisa, parlando di obbligo di formazione: qui stiamo, in realtà, intervenendo sull'obbligo scolastico, che dal 2007 è stato esteso fino a 16 anni con una norma che è richiamata

Con riguardo al primo ordine di problemi, quello riferito alla politica scolastica, vorrei sapere, perché nessuno di noi ha avuto il bene di avere una risposta su questo dal ministro Gelmini, per quale ragione il ministro Sacconi, con l'avallo *ex post* del Ministro dell'istruzione, abbia introdotto questa norma. Gli interpreti della maggioranza del pensiero di Sacconi - e presuppongo anche di quello della Gelmini che questa norma serve per combattere l'abbandono scolastico e cioè per quei ragazzi che a 15 anni non proseguirebbero gli studi Il punto è come si combatte l'abbandono scolastico: uesta norma infatti ha un effetto sul piano della scuola che è quello di deresponsabilizzare completamente la scuola media rispetto all'insuccesso scolastico. Prima di avallare questa operazione, noi dovremmo seriamente interrogarci

precedenti, circa l'anagrafe scolastica, che doveva essere costruita per seguire il successo dei ragazzi e capire perché gli obbligati sfuggano all'obbligo, e quali siano gli interventi di recupero che vengono effettuati.

che le attività laboratoriali sono inutili, che le attività di sostegno non si possono svolgere perché non vi sono più né gli insegnanti né i fondi per pagarli, che le attività *extra* scolastiche sono un lusso che non possiamo più permetterci,

perché essa è sbagliata pedagogicamente e politicamente. In un momento in cui l'Unione europea, e persino la Banca d'Italia, ci richiamano a innalzare i livelli di istruzione dei nostri ragazzi, noi, invece di introdurre norme in positivo per stimolare l'innalzamento dell'obbligo e dei livelli di istruzione e di formazione, introduciamo una norma che sposta in altra sede il problema.

concettuale (non so se sia voluta o meno) tra obbligo scolastico e diritto-dovere alla formazione. Io voglio solo ricordare che non il Governo di centrosinistra, ma quello ancora precedente, ministro Gelmini e anche quello di centrosinistra hanno sottoscritto accordi con tutte le Regioni per dire che il triennio di obbligo formativo - che è diverso, senatrice Maraventano, dall'obbligo scolastico

Ciò ha spostato ancora più in là il concetto di apprendistato, a dopo i 18 anni. Noi lo riportiamo così indietro da fissarlo a 15 anni, senza nemmeno scrivere che è necessaria la licenza media ed avendo contro tutte le categorie

che venga approvato l'ordine del giorno e che si rinvii l'esecuzione del provvedimento per avere il tempo di ragionare sui profili formativi che vogliamo dare a questi ragazzi i quali, proprio perché conseguono un insuccesso scolastico, dovrebbero ricevere la maggiore attenzione

tutta la Commissione sanità, che in modo concorde ha ritenuto, in quel momento, di trovare delle sinergie e far sì che in Aula fosse approvato un provvedimento atteso da lunghissimo tempo. Sia pur minimale, probabilmente, nel suo effetto nell'ambito delle attenzioni al pubblico impiego, esso è importante soprattutto per ritrovare sinergie tra il mondo universitario sanitario e quello degli ospedalieri. L'idea di una sinergia funzionale, oltre quella strutturale che si trova tante volte nelle attività riguardo all'assistenza, è diventata un fatto importante con la norma che oggi trova il suo percorso, così voglio augurarmi, Certo, intervenire sull'età pensionabile per equiparare i medici ospedalieri e i medici universitari non è il massimo dei passaggi culturali che possono produrre effetti significativi in questo settore. Teniamo presente che esistono ancora società scientifiche che vietano, agli universitari e gli universitari agli ospedalieri, di far parte della medesima società scientifica. Ritengo che questo non aiuti a comprendere la propria attività, il proprio sforzo di lavoro, l'intento comune nel favore del paziente. Probabilmente però con questa norma, che oggi trova la sua conclusione nell'ambito del Senato, noi compiamo un ulteriore passo avanti. Diamo cioè uno stimolo a far comprendere che non tanto

che talvolta queste diatribe non hanno altra forza che la conservazione dei privilegi. Allora, il Senato si sforza di rendere operativa in termini concreti questa sinergia importante. È quindi un contributo, anche come spazio culturale, nuovo, di dibattito, di capacità di lavoro comune, che si introduce con questa norma. Dovremmo rappresentare i medici ospedalieri e i medici universitari

di questo tipo? Non credo, però su questa rivendicazione il Parlamento ha posto notevole sensibilità e notevole attenzione. Teniamo presente che nell'altro ramo del Parlamento nel disegno

È una norma che va contro i giovani? È una norma che salvaguarda aspetti particolari? No, anzi. Questa norma per la mia generazione potrebbe non servire, perché noi già a 24-25 anni, appena laureati, anche senza la specializzazione potevamo entrare in ospedale e avere i requisiti per poter raccogliere

maturità professionale. Il chirurgo dopo la specializzazione ha bisogno di altri 10 anni per arrivare ad una completezza di professionalità e di massima espressione del suo lavoro. Allora, avere la possibilità in quel momento di portare il massimo frutto della propria professionalità ritengo sia importante. È un'attenzione che quindi non va

conclude prima di questa norma i 40 anni di servizio effettivo. Invece, diamo lo spazio ai cosiddetti secondari di allora, a quelli che erano gli aiuti e agli altri che, oltre alla beffa talvolta di non poter arrivare ad avere il titolo primariale, avevano anche la beffa di dover essere cacciati prima e di dover andare in pensione. Il primario più anziano poteva rimanere; il giovane aiuto, bravo e altro, doveva andare a casa. uno spazio importante. Ritengo quindi che l'articolo 22, come modificato, per tutti i dirigenti dell'ambito sanitario, non solo per i medici, quindi in modo positivo secondo l'emendamento proposto alla Camera, conceda la disponibilità di avere una permanenza della propria professionalità molto importante e molto qualificata, al di là del titolo che si è raggiunto. Qual è il limite? Il raccordo con l'articolo 72 del perché prevede quella rottamazione possibile da parte delle ASL anche per coloro che con questa norma raggiungono il limite dell'età pensionabile dopo i 65 anni.

del PdL possano apporre la loro firma a quella dei colleghi che hanno proposto quel momento di attenzione per un raccordo assolutamente indispensabile. altro dato che di cui vorrei che il dibattito in Aula conservasse traccia, così come è avvenuto anche in Commissione sanità. Stiamo attenti: nel momento in cui lo abbiamo emendato per la prima volta nel passaggio qui in Aula,

Certo è che, così come emendato anche dalla Camera in questo momento, ritorna e rimane salva la possibilità per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione di poter chiedere alla fine dell'età pensionabile anche i due anni che sono in quel caso a discrezione dell'amministrazione. Ma è una possibilità che naturalmente, pur togliendo quell'inciso, rimane pienamente valida. Noi riteniamo quindi che sia un percorso importante, un'aggiunta significativa verso il raggiungimento della parità tra universitari ed ospedalieri ed ospedalieri che formalmente già raggiungiamo oggi, prima di quello che col disegno di legge sul governo clinico potrà raggiungere la Camera o anche la nostra Assemblea. Vi è una possibilità importante, un aiuto, un passo importante che questo Parlamento offre per far sì che vi sia una coesione maggiore nell'universo sanitario per migliorare l'assistenza. Questa è l'unica finalità. La migliore utilizzazione delle professionalità, la loro maturità piena con la possibilità, insieme agli universitari, alla capacità professionale massima che si è potuta raggiungere, di poterla offrire ai pazienti con serenità, senza nessuna spada di Damocle. Ritengo che questo sia stato un intervento appropriato. Ringraziamo per intero l'Aula, il Parlamento, il Governo per la sensibilità dimostrata nell'accogliere quell'emendamento in quel momento, e poi alla Camera, e per far sì che da quest'oggi si possa naturalmente operare, trasmettendo un ulteriore segnale ed una ulteriore spinta da quest'Aula al mondo universitario ed ospedaliero,

Per la prima volta, dopo tantissimi anni, il Parlamento approva questa norma in favore del comparto sicurezza e del comparto difesa allargato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dove si riconosce la specificità dell'ordinamento, cioè il regime normativo attribuito alle fonti primarie del nostro ordinamento. Dall'approvazione di questa norma conseguirà che le prossime leggi finanziarie dovranno tener conto delle attribuzioni, delle funzioni specifiche del comparto sicurezza e difesa e conseguentemente per la prima volta nella storia del pubblico impiego questo personale dovrà ottenere riconoscimenti normativi ed anche retributivi relativi alle prestazioni aggiuntive che svolgono nelle attività professionali, non ultimo lo vorrei qui ricordare - il rischio della vita che caratterizza le missioni delle Forze armate e delle Forze di polizia all'interno del territorio nazionale. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco vede riconosciuta in questa norma la sua natura di corpo speciale dello Stato ed in forza delle precedenti leggi rinnoverà i contratti collettivi di lavoro nel contesto, appunto, delle risorse che il Governo attribuirà alle Forze armate e alle Forze di polizia. Questa è una rivendicazione

La seconda disposizione su cui volevo soffermarmi riguarda il trattamento per i decessi da amianto, in particolare per il personale militare imbarcato sul naviglio di Stato. Il Governo e la maggioranza dovranno impegnarsi su tale fronte per riconoscere a questo personale i trattamenti che esso stesso rivendica, ma, indipendentemente da tutto ciò, credo che occorrerà snellire le procedure di riconoscimento degli equi indennizzi e delle pensioni privilegiate. Si registra un ritardo di diversi anni sul riconoscimento di queste patologie che trovano origine e causa nel servizio militare e nel servizio di polizia.

del riconoscimento della specificità per il comparto sicurezza e il comparto difesa. Naturalmente è un grande onore per me oggi essere il relatore di questa legge e portare a casa un risultato storico per il comparto sicurezza e difesa. In conclusione, desidero ringraziare tutti coloro, colleghi di opposizione e di maggioranza, che hanno contribuito alla realizzazione di questo obiettivo. Non citerò nessuno, ma credo che questa norma, all'interno di questa legge, sia stata il frutto di una convergenza tra maggioranza e opposizione che riconosce, per la prima volta nella storia, questo principio. PRESIDENTE.

due rapide osservazioni d'impianto in ordine ai temi sollevati, che sostanzialmente si coagulano, da un lato, intorno all'apprendistato, così come novellato dall'articolo 48 e, dall'altro, sul ricorso esteso ed intensificato alla conciliazione e all'arbitrato. Lo dico in particolare agli amici dell'Italia dei Valori, i quali hanno voluto riproporre un'argomentazione che è già comparsa oggi sulla prima pagina di un noto quotidiano e che assumerebbe nella valorizzazione della conciliazione e dell'arbitrato un tentativo di eludere le protezioni di cui all'articolo 18. Mi sembra davvero improponibile un'argomentazione secondo la quale la valorizzazione di un istituto radicato in tutte le migliori democrazie industriali dell'Occidente possa rappresentare un tentativo fraudolento di superamento di un sistema di guarentigie nel quale invece ribaditamente crediamo. Si tratta anzi proprio in questa congiuntura, dopo la grande crisi, di valorizzare l'autonomia delle parti sociali dalle quali promana la regolazione dell'arbitrato e della conciliazione. Conciliazione e arbitrato sono strumentazioni endosindacali tutte le volte nelle quali si ricorre ad esse si affianca alla tutela giurisdizionale classica una tutela che significativamente intensifica la qualità della coesione sociale. È un arricchimento della prospettiva della coesione sociale; è la dotazione di una cassetta degli attrezzi arricchita quella con la quale abbiamo a che fare: altro che tentativo di eludere il sistema dell'articolo 18. Mi ricorda in qualche modo un'osservazione che era stata fatta proprio in Commissione, con la quale venivamo accusati di ribadire l'esistenza di un interesse oggettivo dell'impresa. Noi crediamo profondamente nell'esistenza di un interesse oggettivo dell'impresa, proprio perché a derive liberiste non abbiamo mai acceduto. Crediamo significativamente e densamente alla scansione dell'articolo 41 della Costituzione ed alla vocazione sociale dell'esercizio dello stesso diritto di proprietà. La nostra scuola culturale, la nostra matrice valoriale è quella dell'economia sociale di mercato. Per effetto di questo è ovvio che esista e che sia superiore e distinto rispetto agli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro l'interesse oggettivo dell'impresa come organismo. Altro che affievolimento, altro che indebolimento delle tutele: miglior vocazione, migliore finalizzazione, teleologismo delle tutele. Un ragionamento analogo, illustri colleghi, mi sento di fare per quel che riguarda la contestata norma sull'apprendistato. Ho l'impressione, lo dico in modo molto amichevole e sommesso, che in qualche modo essa si muova da una sopravvalutazione di un impianto dogmatico che è adatto al modello dell'apprendistato del 1955. Con la legge Biagi l'apprendistato, così come lo abbiamo introiettato nella nostra struttura culturale, non esiste più; esistono tre apprendistati significativamente diversi uno dall'altro. In particolare, quello cui mettiamo mano, vale a dire quello funzionale all'espletamento del dovere di istruzione, assomiglia assai poco alla classica configurazione dell'istituto. Siccome nulla incide sulla permanente e ribadita vigenza dell'obbligo scolastico salito a 16 anni, si tratta molto banalmente laddove, al Nord, ad esempio, esista un eccesso di attrattività del mercato del lavoro o, al Sud, un difetto di attrattività della scuola - di riuscire ad intercettare un *drop out* ed a ricondurlo dentro un percorso regolare regolare di convergenza con il mondo misto dell'apprendistato, che assume il ragazzo da una condizione di opacità, spesso di illegalità, per riportarlo dentro un veicolo democraticamente consolidato; ebbene, ciò sarà un grande successo. Quindi, l'unico *driver* di questo provvedimento è la coesione sociale. Crediamo, per una serie di interventi deliberatamente plurali, di aver costruito un sistema nella cui complessità risiede la copertura di zone di gracilità e di fragilità del sistema. Siamo anche disponibili a rimettere mano a tutti questi sistemi, proprio perché non disponiamo di un'algida architettura neoclassica, ma abbiamo la ruvidità, in qualche modo l'impetuosità,

in prospettive di lavoro comune. Crediamo - lo ha ribadito il ministro Sacconi - che dopo le elezioni di marzo, proprio sul territorio del lavoro e della promozione dell'impresa si potrebbero raggiungere intese le quali potrebbero dischiudere una capacità di recupero competitivo del nostro Paese tale non soltanto da traghettarlo oltre la crisi, ma da riportarlo in quella aristocrazia industriale alla quale non può non appartenere. *(Applausi

ribadire alcune valutazioni già egregiamente espresse dai relatori e per aggiungere rapidissimamente qualche considerazione conclusiva rispetto all'*iter* di un provvedimento importante e significativo,

per l'importanza delle questioni che affronta, dei temi che focalizza, dell'itinerario che apre, del processo significativo e importante che mette in moto. Sicché mi soffermerò soltanto sulla parte conclusiva, cioè su quello che nel passaggio tra Camera e Senato si è determinato di sostanzialmente nuovo e rispetto al quale il Senato ha espresso le sue riflessioni e le sue valutazioni. Mi riferisco in particolare al tema dell'apprendistato. Su tale questione, però, mi consentirete, prima di fare le mie considerazioni, di recuperare una riflessione che il relatore, il senatore Castro, ha da ultimo

di sentire un impulso civico prima ancora che politico per fronteggiare alcune questioni laceranti dal punto di vista dell'impatto sociale, ad iniziare dalla questione della dispersione scolastica e della perdita di capitale umano

è intrisa di cultura della sussidiarietà, è spinta sul terreno della bilateralità e della rivalutazione del ruolo e della funzione delle parti sociali rispetto alle novità che sono state introdotte, si spinge sul terreno della cultura partecipativa dove si incrociano diverse storie e diverse culture politiche. Per che è solo un modo per recuperare una sorta di individualismo del lavoratore rispetto al padrone capitalista significa non aver compreso che siamo ben al di là delle culture novecentesche, nel tentativo di affrontare su terreni di nuove sintesi i problemi che abbiamo di fronte. Certo non è con l'approccio ideologico che si risolve il problema della solitudine del lavoratore, del disoccupato e dell'inoccupato, ma a quella solitudine si risponde individuando servizi, provando finalmente a riformare e di cambiare il mercato del lavoro, cercando con il privato, con il privato sociale e con il pubblico di creare i luoghi dove questa solitudine può trovare una risposta, tentando di recuperare in una dimensione nuova e diversa il ruolo, la rappresentatività e la funzione del sindacato. Significa, insomma, rimettere in moto una mobilitazione di carattere sociale che, dentro un quadro di coesione, recuperi il protagonismo delle parti e che sia finalizzata a dare una risposta che non sia quella che abbiamo dietro le nostre spalle. spalle. Anche la riflessione sull'apprendistato si inserisce dentro questa dinamica. Si tratta di uno sforzo, di un tentativo non di abbassare la soglia dell'obbligo scolastico ma di riconoscere una funzione fondamentale al lavoro, per dare risposte attraverso non una norma ma un impulso in direzione della ripresa della riflessione con le Regioni e con le parti sociali per recuperare il valore e l'importanza dell'apprendistato, anche di quello che nella legge Biagi, in Biagi, in relazione all'atteggiamento che non sempre le Regioni hanno assecondato in direzione positiva, non ha trovato il modo di poter esplicitare tutta la sua potenzialità. Noi oggi lo recuperiamo tentando di inserire in un circuito positivo e virtuoso chi lascia il mondo della scuola, della scuola, un circuito quindi che non vuole abbassare il livello ma che cerca di costruire un sistema ed una filiera di cui questo Paese ha bisogno e necessità.

anche aspro in alcune circostanze ma sicuramente utile per cercare di rendere attraverso questo provvedimento il miglior servizio all'obiettivo comune. Tale obiettivo di risolvere alcuni nodi strutturali del nostro sistema per rilanciare il mercato del lavoro, per garantire tutele moderne e per riordinare alcuni sistemi che vanno orientati in maniera positiva al fine di affrontare il tema della filiera dell'istruzione e formazione lavoro, che è la grande questione che abbiamo di fronte.

«La 1a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo». parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, osservando che dalla modifica contenuta nell'articolo 31, comma 8, volta a recepire nella pubblica amministrazione la risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro, potrebbero determinarsi effetti finanziari negativi.

con l'emendamento 1.2 riteniamo che, se da un lato è positivo il fatto che si dia finalmente attuazione alla delega sui lavori usuranti, prevista ormai quasi tre anni fa dal Governo Prodi, non possono non essere rilevate forti perplessità in merito ai meccanismi di priorità nella liquidazione dei trattamenti pensionistici previsti, connessi alla clausola di salvaguardia contenuta al comma 2. Il meccanismo di priorità va infatti garantito in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e a parità degli stessi dalla data di presentazione della domanda. Ciò potrebbe comportare che anche chi abbia maturato i requisiti agevolati potrebbe non vedersi riconosciuto il trattamento pensionistico perché, per una mera questione di presentazione della domanda, potrebbe trovare le risorse esaurite.

il diritto al beneficio rimane condizionato alle disponibilità di bilancio, quindi si tratta non di un diritto assoluto, come dovrebbe essere, ma di un diritto relativo ciò accade sempre quando sono in discussione i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Inoltre il diritto al beneficio dipende, in ordine di priorità, dalla data di presentazione della domanda; dovrebbe dipendere - come noi sosteniamo con l'emendamento 1.1 - più ragionevolmente e più logicamente dalla durata dell'attività lavorativa usurante, prevedendo quindi un criterio oggettivo anziché un criterio burocratico. Per questa ragione chiediamo di votare a favore del nostro emendamento.

circostanziate, ma nemmeno finalizzate negli argomenti, chiaramente quindi indirizzate nel loro futuro dispiegarsi rispetto alle indicazioni del Parlamento. Il provvedimento in esame tratta le questioni più diverse e fra queste anche una delega che noi contestiamo, a cui cerchiamo di apportare le modifiche con l'emendamento 2.1 all'articolo 2, per sottrarre da queste ampie deleghe al Governo quelle che riguardano il riordino di enti che oggi fanno riferimento al Ministero della salute. La delega che il Governo deve adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento prevede diversi decreti legislativi che sono volti appunto a riorganizzare enti, istituti e società che sono vigilati dal Ministero della salute. Questa è una delega nemmeno circostanziata rispetto invece alla denominazione degli enti così com'era stata definita alla Camera, che circostanziava quindi le deleghe al Ministero competente. Inoltre la delega prevede la ridefinizione del rapporto di vigilanza sugli stessi enti e istituti vigilati ed anche la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti di enti o istituti che sono sottoposti alla vigilanza del Ministero competente. Allora è evidente come attraverso questo si prefiguri una ingerenza del Ministero che di fatto annulla l'autonomia di questi enti.

la delega contenuta nell'articolo appare eccessivamente ampia. Si parla genericamente di riorganizzazione di enti, istituti e società vigilati, senza indicare quali essi siano. Il rischio è in particolare di limitare l'autonomia dei soggetti deputati all'attività ispettiva in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'emendamento 2.2, da noi presentato, è volto da un lato a salvaguardare la pur giusta necessità di un coordinamento fra i soggetti aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ma dall'altro lato anche a specificare la necessità di rispettare la competenza e l'autonomia di ciascun ente.

**Il Senato non approva.**

l'approvazione della legge sulle missioni all'estero abbiamo approvato - anzi, avete approvato - un emendamento che sottraeva i militari i militari dalle eventuali responsabilità sul terreno del non rispetto della legge sull'amianto e, più in generale, sulla sicurezza del lavoro. Avevate detto che lo Stato si sarebbe fatto carico di questi problemi.

ci troviamo di fronte al fatto che non solo non si colpiscono i responsabili, ma non si danno neanche delle soluzioni ai lavoratori sul naviglio di Stato, che in gran parte sono militari. Questo è estremamente grave. Pensiamo che questo articolo debba essere soppresso, perché lede lavoratori e servitori dello Stato che più di altri si espongono per la sicurezza del nostro Paese, perché, fra l'altro, noi vorremmo che la politica si occupasse di queste cose e non lasciasse solo alla magistratura il compito di dare una giusta soluzione a questi lavoratori. Negli emendamenti seguenti proponiamo delle soluzioni delle soluzioni che almeno diano delle risposte giuridiche ed economiche a questi lavoratori che versano in condizioni economiche

Capisco che voi non approviate niente di questa normativa, sbagliando, come altri miei colleghi hanno detto, ma almeno su questo terreno proviamo a predisporre un ordine del giorno che possa individuare

Troviamo almeno una strada di speranza. Capisco che un ordine del giorno non risolve assolutamente il problema, ma almeno facciamoci carico del fatto che un problema esiste, fermo restando che andrebbe soppresso tutto l'articolo.

dalla data di entrata in vigore di questa legge, un decreto ministeriale al fine di integrare la disciplina di protezione riguardo a questi lavoratori colpiti dagli

In relazione alla riflessione del senatore Nerozzi, manifesto fin d'ora la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno cui

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", premesso che l'articolo 20 del provvedimento reca una interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, con la quale si stabilisce che ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, lettera *b)*, della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito, impegna il Governo, sentiti gli Enti preposti, ad individuare la platea dei lavoratori del naviglio di Stato esposti e le necessarie coperture economiche al fine di valutare gli interventi da assumere. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà. CASSON *(PD)*. Signor Presidente, l'articolo 20 del disegno di legge in esame si pone in netto ed evidente contrasto con le dichiarazioni del Governo e della maggioranza di voler intervenire con questo provvedimento a tutela dei lavoratori. Questo articolo 20 propone una sorta di interpretazione autentica di una vecchissima e consolidata norma posta a tutela dei lavoratori fin dal 1955, norma ripetutamente e pacificamente applicata nel tempo da organi amministrativi, dalla polizia giudiziaria e dalla magistratura, nei rispettivi ambiti di competenza, soprattutto per i casi di infortunio sul lavoro e di malattie professionali. Tanto è vero che, anche di recente, sono stati instaurati dei processi penali a carico delle persone ritenute responsabili, per colpa, della malattia e della morte di lavoratori a causa dell'amianto. E in particolare, davanti all'autorità giudiziaria di Padova è pendente un processo per la morte da amianto di alcuni militari. E altri processi seguiranno, perché sono ormai circa seicento i militari della nostra marina colpiti da patologie asbesto-correlate e non si capisce per quale motivo i nostri militari non dovrebbero essere tutelati dalle malattie professionali. In questo momento, con questa norma, con una piroetta giuridica, nel tentativo di dare una mano ai responsabili di vertice (secondo l'accusa) di quei decessi e di sottrarli ai processi e all'eventuale condanna, si vorrebbe cambiare la legge, secondo uno stile deplorevole e vergognoso già visto in altre occasioni e che sembra caratterizzare il modo di pensare e di agire di questo Governo e di questa maggioranza. Una legge non va bene? C'è il rischio di un processo e di una condanna penale? La soluzione è a portata di mano, per il Governo. Un colpo di spugna e via. Il giochino perverso è molto semplice: si cambia la legge, infischiandosene dei profili di illegittimità costituzionale e del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. E nel caso di norme già contestate agli imputati e applicate dalla magistratura, si fa come in questo caso: la norma va interpretata, autenticamente, come dice questo Governo e non come logicamente e correttamente farebbe qualsiasi persona normale, di buon senso, qualsiasi interprete del diritto, con ciò tentando di salvare qualcuno ai vertici militari, a discapito di altri militari di grado inferiore deceduti solo per aver fatto il proprio dovere. È, questa dell'articolo 20, una manovra viscida e vergognosa, perché nascosta nelle pieghe poco comprensibili di commi e contro-commi. E soprattutto è paradossale, perché si pone all'interno di un provvedimento che avrebbe come finalità la tutela del lavoro e la sicurezza sul lavoro, anche militare, mentre invece, con un'interpretazione autentica di una legge di 55 anni fa, si determina, deliberatamente, un vuoto normativo proprio in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro. Ha poco senso quanto detto poco fa dal relatore, senatore Saltamartini, che ha detto che il Governo dovrà impegnarsi, che ci sono ritardi di anni e che il tema amianto sarà risolto: intanto i lavoratori muoiono. È pilatesco, è un vero e proprio colpo di spugna, conforme ad una consolidata politica di questo Governo, anche in materia di sicurezza sul lavoro. Signori della maggioranza, decidetevi. I lavoratori non si tutelano soltanto con le parole, ma con i fatti. E nella nostra veste di senatori si tutelano approvando leggi che siano davvero a salvaguardia della loro integrità e dei loro diritti.

dare un segno significativo affinché in questo provvedimento ci sia, effettivamente, la volontà di migliorare le condizioni di lavoro e di partecipazione delle donne. così non sembra. È noto che noi siamo contrari alla scelta di dilazione dei termini per l'approvazione della delega e al superamento dei Comitati per le pari opportunità contenuti nella legge n. 125 del 1991 (superamento intervenuto con le modifiche dello scorso passaggio al Senato, che li sostituiscono con dei generici comitati antidiscriminatori e per il benessere). Io voglio richiamare, con questo ordine del giorno, l'attenzione alla necessità di rafforzare, ora e subito, le iniziative per sostenere l'effettiva promozione delle pari opportunità e della partecipazione delle donne al lavoro. Abbiamo già richiamato moltissime volte, in quest'Aula, la condizione delle donne in questo Paese e non sto, quindi, a ricordarla. È noto a tutti quale sia la situazione, rispetto agli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona, rispetto ai divari reddituali e rispetto alla rappresentanza nella classe dirigente e in politica. Vi chiedo di impegnarci tutti per superare questo *gap*. Abbiamo l'occasione per farlo, in quanto sono incardinati al Senato diversi disegni di legge in materia di partecipazione delle donne al lavoro e di rappresentanza. Ve ne sono poi altri, presentati sia alla Camera che al Senato, che ragionano in materia di diritti di partecipazione delle donne alla *governance* delle imprese, con particolare riferimento alle società quotate e alle società pubbliche. Quindi, portando avanti rapidamente la discussione su questi provvedimenti, c'è l'occasione, di fare qualcosa di concreto, e di farlo subito, per garantire una migliore partecipazione delle donne al lavoro alla direzione di questo Paese, sia nelle imprese che nella politica. Vi chiedo, pertanto, di esprimere un parere favorevole a questo ordine del giorno.

*relatore*. Signor Presidente, la proposta conclusiva, il punto di caduta, come si dice in gergo negoziale, è quella relativa all'accoglimento dell'ultima fra le premesse,

se l'accoglimento del dispositivo implica, come credo sia già stato proposto in sede di Ufficio di Presidenza, una corsia accelerata per il provvedimento sul lavoro che abbiamo in Commissione, sono disponibile ad accogliere la riformulazione.

di legge di cui abbiamo discusso in apertura di questa seduta: la questione dell'arbitrabilità delle controversie in materia di impiego pubblico. ricordare, proprio a proposito dell'ordine del giorno menzionato adesso dal collega Castro, che ieri in Commissione...

un ordine del giorno che impegna il Governo stesso a emanare disposizioni affinché l'arbitrato che con la norma al nostro autorizzare nelle controversie di impiego pubblico non venga attivato dalle amministrazioni. Ne consegue che stiamo per votare una norma

chiesto che venga respinto l'emendamento soppressivo di questa norma.

Signor Presidente, al comma 9 dell'articolo 31, riguardante le modalità di espletamento dell'arbitrato, afferma che, in assenza di accordi sindacali, categoriali o confederali, e trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge (quindi in mancanza di accordo sindacale

Per noi è del tutto evidente che non basta (questo è il punto) una semplice consultazione sindacale per evitare la possibilità di aggirare l'articolo 18 Per questa ragione, con l'emendamento 31.6 chiediamo che si proceda (questa è la modifica che l'emendamento propone) «d'intesa» con le parti sociali. Non è un problema formale o lessicale, ma è una questione sostanziale, perché solamente con il vincolo dell'intesa con le parti sociali si può

non sono voluto intervenire prima di adesso, ma vorrei fare un breve ragionamento per ripercorrere questa vicenda che è da più di un anno che si trascina, anche per altri versi, ma su questo punto in particolare. Noi abbiamo sempre denunciato che questa norma è pericolosa e addirittura sovversiva in senso tecnico di tutto il diritto del lavoro.

non contino, oppure che possano essere violati i limiti massimi di orario di lavoro o che le norme sulla sicurezza siano un *optional*. Evidentemente questi sono casi estremi, ma se un arbitro è libero, cioè non ha il vincolo del rispetto delle norme inderogabili di legge, può succedere anche questo, senza possibilità che si ricorra al giudice. un tipo di arbitrato del genere non esiste da nessuna parte, neanche negli ordinamenti più liberisti. Io ho frequentato a lungo lungo gli Stati Uniti e l'Inghilterra ed anche gli arbitri di quei Paesi (che, tra l'altro, sono anche professori universitari, quindi è un mestiere che potrebbe essere interessante) e siamo favorevoli all'arbitrato, lo abbiamo detto più volte, ed anche a

le indicazioni dei contratti collettivi può essere assolutamente utile, anzi, avevamo anche detto che le parti dei contratti collettivi, siccome hanno creato dei diritti propri,

Tale norma avrebbe avuto il vantaggio di dare all'arbitro un largo spazio di manovra, che adesso non c'è e a me dispiace perché sono anni che diciamo che vorremmo che tale istituto venisse utilizzato di più. Ma una cosa è dire questo, altro è che l'arbitro può decidere anche senza rispettare le norme inderogabili del diritto del lavoro. Il richiamo presente nel testo ai principi generali del diritto è comunque utile ma

senza la protezione storica del diritto di lavoro, bene, si affrontino - come si è già fatto, del resto - le singole norme e si dica, ad esempio: «Questa norma è troppo rigida, la rendiamo più morbida, la deregoliamo». È successo

delle norme del diritto del lavoro. Questo è assolutamente inaccettabile. L'altro argomento che si avanza è: il lavoratore, in fondo, non è così un poveretto. Beh, no, non è un poveretto, però tutto il diritto del lavoro, almeno nei suoi aspetti fondamentali, è nato sul presupposto

è incredibile che in un sistema che non ha mai usato l'arbitrato, perché c'è un eccessiva diffidenza, a mio avviso, nei suoi confronti, adesso si passi da un uso nullo dell'arbitrato (sbagliato) a un uso selvaggio di tale istituto, che, ripeto, non vedo neanche negli Stati Uniti e nell'Inghilterra, Paesi notoriamente liberisti. Non è accettabile un modo di ragionare così: forse è inconsapevole (ma non credo perché è passato un anno e mezzo), ma è assolutamente devastante devastante per il diritto del lavoro. Notate che i colleghi Ichino e Morando hanno detto che, per quanto riguarda il pubblico impiego, ciò è sicuramente incostituzionale,

all'arbitrato libero nel diritto privato, cioè nel rapporto di lavoro privato, nella quale si prevede che un singolo, da solo e senza l'assistenza dei sindacati, magari sotto assunzione o sotto rinnovo del contratto, può firmare un pezzo di carta in cui c'è scritto che l'arbitro può fare quello che vuole,

credo che anche questo aspetto sia molto opinabile. Per questo motivo abbiamo rivolto appelli reiterati a riconsiderare questa norma e ci sembra un dovere civico fondamentale denunciarla e votare contro

nostro esame non soltanto è il frutto di un intenso lavoro parlamentare durato due anni - siamo alla quarta e mi auguro ultima lettura - ma ma soprattutto ha un'origine che voglio ricordare all'Aula per capire quanto ponderate siano state le considerazioni che hanno condotto a quell'equilibrio. L'autore fu Marco Biagi,

che poi, proprio al Senato, fu stralciato su richiesta delle organizzazioni sindacali di una più attenta considerazione; quella stessa considerazione che poi ha portato alla novità, introdotta nell'ambito del percorso parlamentare, del rinvio alla contrattazione collettiva, o comunque ad una fase di intensa contrattazione collettiva della quale

un linguaggio che per chi come me ha vissuto una certa stagione non può non indurmi a chiedere di contenere le pur legittime critiche che possono essere rivolte a questo testo entro quella moderazione che si consiglia in presenza di terzi che non hanno mai accompagnato civilmente il nostro dibattito,

che l'arbitrato per equità possa significare deroga a norme che, in quanto inderogabili (lo dice la legge stessa), non potrebbero essere certo non tenute in considerazione dall'arbitro ed ipotizzare uno scenario che onestamente non sarebbe nell'ordine delle cose possibili se un domani questo testo venisse approvato. Solo queste riflessioni volevo rimettere all'Aula perché, ripeto, le pur legittime considerazioni e comprensibili critiche da parte dell'opposizione tengano conto di un percorso e tengano conto

sono state coinvolte anche le parti sindacali, e infatti per un percorso si è cercato di ammettere un arbitrato gestito, controllato delle parti sociali, però, non dimentichiamo - e il Ministro lo sa - che c'è un altro pezzo della norma in cui l'arbitrato può essere fatto anche dal singolo, fuori da qualsiasi e percorso contrattuale.

il principio fondamentale della nostra Costituzione e del diritto del lavoro. È chiaro che l'arbitro potrebbe anche comportarsi bene, ma bisogna pure che l'arbitro abbia delle guide. Noi avevamo proposto che l'arbitrato si potesse fare liberamente rispetto alle norme contrattuali, ma non rispetto alle norme di legge: è il modo normale per controllare e prevenire anche abusi in buona fede.

nella norma manca il *dies a quo*, cioè il momento dal quale il termine dovrebbe decorrere. Tale norma, così com'è, genererà soltanto un contenzioso infinito e facilmente evitabile.

non porterà ad una liberalizzazione selvaggia, perché la stragrande maggioranza degli imprenditori italiani

Quindi non ci uniamo al coro di chi dice che qui viene smantellato il diritto al lavoro, ma lamentiamo che questo Governo continua ad intervenire sistematicamente sui lavoratori di serie B e C e magari anche di serie D. È a loro che voi togliete i diritti,

chiedo scusa per non essere stato pronto nella risposta, ma un grande turbamento personale mi ha colto e soltanto il rispetto che porto a quest'Aula mi ingiunge a non dare corso ad un'operazione, che trovo assolutamente impropria, di disappropriazione di una memoria per me personalmente sacra. Constato solo - e non sto parlando di Marco Biagi - che sono state definite faccendieri le organizzazioni sindacali, le università, perché chi può certificare i contratti nell'ambito dei quali può essere attivata la procedura arbitrale sono soltanto i soggetti certificati e, in base alla legge Biagi, i contratti certificati possono essere resi tali solo dalle

Presidente, illustro l'emendamento 46.2 (testo 2). Abbiamo più volte ribadito in quest'Aula che l'attuale crisi economica e le gravi conseguenze che essa ha avuto sul piano occupazionale rende non più rinviabile l'esercizio delle deleghe in materia di ammortizzatori sociali, previsti dal protocollo sul *Welfare*. In quest'ottica gli interventi emendativi proposti sono volti ad accorciare il termine previsto per l'esercizio della delega. La norma in oggetto fissa, infatti, il termine in 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento attualmente in esame. Gli emendamenti che proponiamo indicano, invece, il termine per l'esercizio della delega in 36 mesi a partire dell'entrata in vigore - ovviamente già avvenuta - della legge n. 247 del 2007. Pertanto, con l'approvazione del nostro emendamento, rimarrebbero ancora nove mesi

direzione dell'attuazione della delega sugli ammortizzatori sociali, sulle politiche attive del lavoro, sull'occupazione femminile e che i termini per l'esercizio della medesima siano i più brevi possibile. Tuttavia, il modo in cui si è intervenuti nella dilazione dei termini della delega è, dal punto di

precisando nuovamente che occorre che la delega sia attuata nel più breve tempo possibile e che è inaccettabile questo modo di legiferare, che rende le norme assolutamente incomprensibili e contraddittorie.

non condividiamo l'abbassamento dell'obbligo scolastico da 16 a 15 anni. Ricordo che il prolungamento a 10 anni dell'istruzione obbligatoria è stato introdotto soltanto nel 2006, mentre era già previsto nella maggior parte dei Paesi europei. Un ritorno al passato potrebbe causare un ulteriore aumento del già preoccupante fenomeno dell'abbandono scolastico, che interessa in modo particolare il settore dell'istruzione tecnica e professionale. È un fenomeno grave, che comporta l'abbassamento del livello della qualità di manodopera, in netta controtendenza con le esigenze delle imprese.

La norma, infatti, consente di stipulare un contratto di apprendistato con ragazzi di 15 anni e prevede che questo valga come obbligo dell'istruzione. È una norma a nostro avviso gravissima, con impatti molto pesanti sul piano sociale e su quello economico, in quanto abbassa l'età minima di ingresso nel mondo del lavoro dai 16 ai 15 anni. L'età minima era stata fissata dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 622) a 16 anni, in coerenza con l'innalzamento a 16 anni dell'obbligo di istruzione. «L'istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria», così recita la norma. Ed allora chiedo alla maggioranza e al Governo se ritengono accettabile oggi, nel 2010, abbassare l'età di ingresso nel mondo del lavoro;

Non è accettabile, rappresentante del Governo, che su questo tema valga la logica del male minore; così come non è accettabile che si risponda all'abbandono scolastico dicendo che è meglio che i ragazzi vadano a lavorare il più presto possibile se non sono capaci di stare a scuola. L'unica reale risposta all'abbandono scolastico è quello di contrastarlo e di farlo attraverso investimenti adeguati sulla scuola media e sui primi anni della scuola superiore, su cui si concentrano in particolare gli abbandoni scolastici. Lo si deve fare con investimenti nei laboratori, nell'innovazione, nelle esperienze scuola-extra scuola, scuola, nelle esperienze di *stage* e anche di alternanza scuola-lavoro. Certamente, tutto il contrario di quello che sta realizzando oggi il ministro Gelmini ed io chiedo al sottosegretario Viespoli di non confondere, come viene fatto e come è stato fatto in quest'Aula, il ruolo dell'alternanza scuola-lavoro, dello *stage* e dei percorsi di esperienze lavorative dentro la scuola o all'interno della formazione professionale, con il contratto di apprendistato. L'apprendistato non è un percorso di istruzione, è un contratto di lavoro, mentre *stage* alternanza scuola-lavoro ad esperienze lavorative si situano all'interno di percorsi scolastici e formativi, perché volti all'apprendimento e accompagnati da docenti, *tutor* e da personale educativo. È questa la differenza sostanziale, mentre l'apprendistato è un puro e semplice contratto di lavoro. Lascio immaginare a tutti i senatori come può essere qualificato e come può essere formativo un contratto di lavoro fatto per un ragazzino di 15 anni, debole sicuramente, emarginato, che ha abbandonato la scuola, che non ha neanche, in alcuni casi, la terza media e che probabilmente a stento sa leggere e scrivere. Voglio ricordare che anche nel contratto di apprendistato formativo cui si fa riferimento in questa norma, (quello che deve essere applicato ai minori di 18 anni) le ore di formazione sono 240. 240. Raffrontiamo queste 240 ore con le 800, 900 o 1.000 che corrispondono invece ad un percorso di carattere scolastico. Voglio ricordare - anche questi sono dati dell'ISFOL - che nel 2007 solo 6.500 ragazzi (meno del 20 per cento dei ragazzi minori che fanno apprendistato) hanno potuto usufruire di una formazione esterna alle imprese. Quindi, ci troviamo di fronte a una norma

Chiedo al Senato di essere molto consapevole, molto responsabile e molto attento su questa scelta, perché spetta a noi decidere, ovviamente ignorando la vulgata popolare secondo la quale chi non ha voglia di studiare è bene che vada a lavorare molto presto, soffermandosi invece sugli effetti reali di questa norma: riducendo di un anno l'investimento nell'istruzione si ridurranno le opportunità di futuro dei ragazzi, soprattutto di quelli più deboli e in difficoltà; si abbasserà ancora la bassissima mobilità sociale che c'è in questo Paese, per cui sempre più chi ha dei genitori formati e che hanno una buona professione avrà un'opportunità di lavoro, mentre tutti gli altri saranno esclusi: si bloccherà ancora di più la mobilità sociale. Si ridurrà la possibilità di sviluppo economico, occupazionale e di prodotto interno lordo perché, come ci hanno autorevolmente mostrato importanti indagini dell'OCSE e recenti studi della Banca d'Italia, un innalzamento di un anno dell'istruzione obbligatoria

poiché già in Commissione il Governo ha espresso parere negativo sull'emendamento 48.8 che riguarda gli *stage*, chiedo al ministro Sacconi, poiché in Italia

ha intenzione di affrontare questa questione o ritiene che questa parte del mercato del lavoro debba essere abbandonata a sé stessa, nonostante quanto accade sotto i nostri occhi quotidianamente.

tra i quali quello di aumentare il numero dei diplomati. Il ministro Moratti aveva messo molto chiaramente tra i suoi obiettivi il diritto-dovere molto più realisticamente il Governo Prodi aveva inserito nella finanziaria 2007 l'obbligo all'istruzione fino a 16 anni di età, con l'inserimento nel mondo del lavoro a 16 anni. obbligo all'istruzione che favoriva la formazione professionale triennale, quella più seria che ad esempio i colleghi della Lega Nord dovrebbero conoscere bene, come quella della Lombardia e del Veneto, che viene messa in crisi da questo provvedimento. Attraverso quella formazione professionale triennale si permetteva agli alunni che non avevano ottenuto la licenza media di recuperarla. Ora, con questo provvedimento si consente ad un ragazzo di 15 anni che non ha la terza media di affrontare il mondo del lavoro con un contratto di apprendistato,

un sistema di autorizzazioni alle aziende, di definizione delle qualifiche e dei requisiti per i *tutor* come già vigenti in alcune Province autonome del nostro Paese; il requisito minimo del diploma di scuola secondaria di primo grado, perché non sarà più recuperabile in altro modo. Quando infatti si è detto che i ragazzi poco motivati dalla scuola saranno comunque recuperati dalla strada, mi domando: per quanto tempo, con lavori precari, con scarsa preparazione, con nessuna professionalità?

*(PdL)*. Signor Presidente, solo per completezza di informazione, in riferimento all'intervento della senatrice Bastico, che ha citato correttamente lo studio della Banca d'Italia, devo precisare che nello studio della Banca d'Italia si dimostra che il rendimento più alto si ottiene dall'investimento in istruzione con una media del 7 per cento; ma nello stesso studio si dice che per ottenere quel risultato occorre anche tener conto della dispersione e cioè della meritocrazia, cioè della istruzione in base al merito. L'intervento sul piano sociale, quindi, semmai va fatto *ex ante*, nelle fasce iniziali dell'istruzione

sul lavoro, si dimostra che, piuttosto che disperdere anni inutili in una formazione scolastica a rendimento zero

mi è venuto spontaneo chiedere di parlare brevemente, a causa del tempo contingentato, dopo l'intervento del professor Baldassarri. Un professore, cioè una persona che deve avere a cuore sommamente di rimediare e, come la nostra Costituzione richiede, di rimuovere gli ostacoli.

Siccome il senatore Castro ha parlato di complessità e io seguo il suo ragionamento, se noi avremo lavoratori ignoranti, essi non parteciperanno ai processi di innovazione. Noi abbiamo bisogno di chi, lavorando, sappia anche come lavorare e non è quella l'età in cui si possano apprendere, oltre alle manualità, anche le competenze intellettuali. A noi sembra che questo sia stato uno scivolone.

Signor Presidente, in tanta animata discussione credo che qualche volta si finisca per assumere posizioni assolutamente inconciliabili in maniera definitiva, mentre si dovrebbe avere a cuore l'interesse dei giovani ai quali facciamo riferimento. Vorrei ricordare alla collega Mariapia Garavaglia che c'era anche un'altra persona molto attenta ai problemi del disagio giovanile, soprattutto in una fascia particolare quella quale quella degli adolescenti: si chiamava Don Bosco. Il sistema preventivo dell'educazione, soprattutto nei confronti dei ragazzi che avevano particolari difficoltà di inserimento nella scuola e un rendimento scolastico bassissimo, prevedeva l'avviamento ad

di recuperare questo svantaggio culturale tempestivamente, attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro, che non deve essere il lavoro forzato, ma un lavoro altamente e profondamente educativo. Si può fare educazione professionale

Il massimo dei punti d'incontro praticabile è già stato consolidato in Commissione con l'ordine del giorno approvato in quella sede.

48 proprio perché contiene la norma di cui ha parlato la senatrice Bastico prima: quella che prevede che l'obbligo di istruzione possa essere assolto nell'apprendistato. Per noi questa è una norma inaccettabile, regressiva e punitiva. Diciamo che è un atto di leggerezza, di grande leggerezza da parte del Governo e della maggioranza verso i giovani. È regressiva perché fa tornare indietro la legge vigente, è regressiva rispetto agli obiettivi che ci pone l'Europa, la quale ci chiede di fornire più istruzione obbligatoria e non meno istruzione; ci chiede di ridurre la dispersione scolastica, di aumentare il numero dei diplomati. Quando abbiamo chiesto in Commissione

consentiamo che sulla loro testa si facciano contratti di lavoro al di fuori di ogni percorso formativo, a 15 anni. Chi li accompagnerà nell'apprendistato? Chi si prenderà cura di questi ragazzi ? Nessuno. Saranno abbandonati a loro stessi.

si dovrebbe chiedere perché non hanno voglia di studiare, come rimediarvi, come rendere la scuola più interessante anche per quegli studenti che sono più restii allo studio. Certo, colleghi, lo so che è più facile la scorciatoia della deresponsabilizzazione della scuola. Sicuramente si risparmia, ed è ciò che voi volete e che vuole il ministro Tremonti: infatti ci sono sempre meno insegnanti nella scuola, meno insegnanti di sostegno; sempre più difficile il contatto tra docente e studenti; classi sempre più numerose. State creando una scuola che esclude e non che include. Siete molto lontani da quella scuola del «non uno di meno» che noi vogliamo. Certo: il sapere è anche saper fare, manualità, creatività individuale, ma c'è una tradizione pedagogica di prima grandezza nel nostro Paese basata sull'apprendimento attraverso l'attività dei laboratori. Valorizziamo quella attraverso la sperimentazione, ma restiamo dentro il percorso di istruzione. Voi fate una perniciosa confusione tra istruzione, formazione e, per di più, Non sono la stessa cosa, colleghi; l'ho detto in Commissione e lo voglio ripetere in Aula: è l'istruzione che dà gli strumenti per imparare ad imparare e continuare a farlo lungo tutto l'arco della vita, per affrontare il lavoro flessibile, per sviluppare la capacità di aggiornarsi, di imparare una lingua ad usare le nuove tecnologie. Senza questi strumenti minimi si creano degli emarginati sociali. salire dopo questo vostro provvedimento il numero di coloro che non riusciranno ad integrarsi nel mondo del lavoro: altro che coesione sociale, senatore Castro. Allora noi votiamo no, perché non vogliamo e non tolleriamo che i nostri ragazzi paghino lo scotto della vostra miopia, della vostra leggerezza e della vostra irresponsabilità.

il testo del presente disegno di legge ci ha consentito di approdare a soluzioni condivisibili su diversi temi, anche per la disponibilità da parte della maggioranza e del Governo. Altri aspetti rimangono critici. Quella che stiamo affrontando oggi è una battaglia di civiltà - una civiltà che nel dibattito è sembrata quasi sparire al fine di riconoscere finalmente a tutti quei lavoratori esposti ad attività faticose e usuranti un trattamento migliore e dunque poter accedere alla pensione in maniera anticipata, considerata la peculiarità dei lavori e il rischio per la salute di questi ultimi.

sappiamo, che purtroppo dalla prima lettura, che risale a due anni fa, fino ad oggi, le problematiche del nostro Paese a livello di precariato non sono diminuite ma aumentate. L'occupazione è peggiorata gravemente, viviamo un momento di crisi; sarebbe pertanto urgente e necessario che le misure sugli ammortizzatori sociali fossero attuate con urgenza e non con questa dilatazione di termini che purtroppo abbiamo approvato nell'articolato. Sono state approvate alcune proposte parlamentari che apprezziamo, quali il ripristino della gratuità per i processi sul lavoro e le norme per i Vigili del fuoco.

che un peso burocratico e sanzioni su tutte le aziende italiane, piccole e medie, che stanno soffrendo questo momento di crisi. Sulla questione delle trattative si sarebbe dovuto discutere un po' di più. Sono d'accordo che non si debba abbassare il limite della protezione dei lavoratori,

(l'ex ministro senatore Treu lo sa perché ci ha dato una mano) nell'ambito della previdenza complementare, dove siamo riusciti a costruire un modello veramente di avanguardia e anche di esempio a livello europeo. Per quanto riguarda l'articolo 20 dal momento che la norma introdotta incide sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e pertanto necessita di una più attenta ponderazione. In merito all'articolo 22, rileviamo l'eccessiva confusione e la disorganicità degli interventi da parte del Governo in materia previdenziale. Si è determinata una grande incertezza per i dipendenti pubblici sull'anzianità, anagrafica e contributiva, e sul loro collocamento a riposo su base volontaria o coatta. Quest'ultimo aspetto è grave in quanto la permanenza in quanto la permanenza a servizio del lavoratore è fatta dipendere dall'incondizionata discrezionalità dell'amministrazione di appartenenza. Manifestiamo invece apprezzamento

prevedere un adeguato numero di ore di formazione e un adeguato percorso professionale che sia effettivamente qualificante.

Signor Presidente, colleghi, ci è stato spiegato più volte che il provvedimento che andremo tra breve a votare costituirebbe un semplice e «liberale» passo indietro dello Stato nella logica di un incontro libero tra le forze del lavoro nell'ambito del mercato. Il diritto del lavoro, sin dalla sua nascita, si è basato sul riconoscimento che nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, i due soggetti non possono essere considerati sullo stesso piano perché, oggettivamente, il lavoratore costituisce, rispetto all'impresa, una parte debole e dunque meritevole di maggiore tutela. Al contrario, come abbiamo già avuto occasione di rilevare più volte, siamo in presenza di un provvedimento il cui quadro normativo risulta totalmente sbilanciato a favore del soggetto già di per se forte, cioè l'azienda. Naturalmente tutto ciò rientra coerentemente all'interno di un disegno complessivo portato avanti dal Governo sui temi del lavoro. Anche in questo caso, la maggioranza sembra muoversi su due direttrici ben precise: demolizione delle garanzie dei lavoratori e smantellamento del cosiddetto Protocollo sul *Welfare* del 2007. L'opera di demolizione delle garanzie già esistenti per i lavoratori è qui, come in altri provvedimenti, attuata attraverso l'inserimento di norme che, pur non intervenendo direttamente sulle garanzie in questione, ne intaccano l'efficacia creando spazi normativi per un loro agevole aggiramento. Nel novero di queste ultime norme rientrano sicuramente, ad esempio, le previsioni di cui agli articoli 5 e 7 nonché le modifiche al codice di procedura civile contenute nel famigerato articolo 31. L'articolo 5 riguarda le cosiddette misure contro il lavoro sommerso. Tuttavia, ciò che si comprende, anche da una rapida lettura, è che tra la rubrica e il testo della norma non si riscontra alcuna connessione. Anzitutto, non si comprende perché, visto che l'obiettivo dovrebbe essere contrastare meglio il fenomeno del lavoro sommerso, si ritenga utile stabilire una riduzione delle sanzioni a carico dei datori di lavoro che assumono in maniera irregolare. Assolutamente incomprensibile è la previsione in base alla quale non si applicano le sanzioni collegate alle irregolarità contributive «qualora si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto di lavoro». Vorrei sapere se qualcuno, sinceramente, è in grado di spiegare come si dovrebbe applicare nella pratica una simile formulazione. Sempre a proposito di lavoro sommerso, si prevede inoltre la possibilità di posticipare la comunicazione dei dati del lavoratore sia per il settore turistico (già di per se costantemente interessato da abusi) sia addirittura per il settore del pubblico impiego. Quanto all'articolo 31, esso introduce un vero e proprio arbitrato obbligatorio a pagamento nelle controversie di lavoro. Innovando quanto finora disposto dal codice di procedura civile, si stabilisce che il lodo arbitrale sia impugnabile di fronte alla corte d'appello solo ove ciò sia stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia. Questo appare particolarmente grave se letto in combinato disposto con la previsione dell'obbligatorietà dell'arbitrato.

tratta pertanto di una scelta che va fatta sempre *ex ante*, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro; soprattutto, manca un obbligo, per chiunque, di comunicare al lavoratore che, se vuole conservare la *chance* di rivolgersi alla magistratura, deve scriverlo nero su bianco prima. Veniamo ora alla seconda direttrice dell'azione del provvedimento in esame, cioè alla demolizione delle innovazioni conseguite con il Protocollo sul *Welfare*. Qui l'orientamento che sembra delinearsi è invece un puro e semplice ritorno a quanto previsto dal testo originario del decreto legislativo Abbiamo più volte sottolineato la gravità della decisione di reintrodurre lo *staff leasing*, cancellato con la concorde volontà di tutte le parti sociali nella legislatura precedente. Ora ci troviamo davanti ad una norma sull'apprendistato della cui insensatezza e potenziale dannosità per i giovani e per il loro ingresso nel mondo del lavoro abbiamo già ampiamente parlato. Riteniamo superfluo ritornarvi diffusamente, ma non altrettanto superfluo ribadire la nostra ferma contrarietà ad essa. Resta poi il nodo fondamentale, anche questo già segnalato all'inizio e sul quale abbiamo cercato con i nostri interventi emendativi di apportare quanto più possibile dei miglioramenti, delle deleghe al Governo in materia di lavori usuranti e di ammortizzatori sociali. Per quel che riguarda i primi, purtroppo restano tutti gli aspetti negativi che abbiamo cercato di segnalare nel corso del dibattito. In particolare, ribadiamo le nostre perplessità circa le modalità previste per il riconoscimento dei trattamenti pensionistici e i meccanismi di priorità per la liquidazione degli stessi. Ancora più grave è invece la decisione della maggioranza di confermare il rinvio di altri due anni dell'esercizio della delega degli ammortizzatori sociali. Tale decisione risulta insensata alla luce dei dati forniti dall'ISTAT, che hanno rilevato come il tasso di disoccupazione sia in continua crescita e a gennaio abbia raggiunto l'8,6 per cento. Sempre nel mese di gennaio, il numero delle persone in cerca di occupazione risulterebbe pari a oltre 2 milioni, in crescita del 20 per cento rispetto a gennaio 2009. In questo momento, un provvedimento sul lavoro di questa portata avrebbe potuto costituire un'occasione per approvare norme volte a risolvere davvero i problemi del mondo del lavoro. Dobbiamo invece constatare che, nonostante si stiano avverando le più fosche previsioni riguardo alla situazione occupazionale del nostro Paese,

deciso comunemente di stringere i tempi per le dichiarazioni di voto finale, i colleghi possono consegnare la parte dell'intervento che non riescono a svolgere Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, i motivi per cui sosteniamo questo provvedimento e lo condividiamo sono stati ampiamente illustrati dal mio Gruppo in sede di prima lettura e dalla collega Maraventano in sede di discussione generale.

suo contenuto. Questo disegno di legge costituisce probabilmente la manifestazione più clamorosa della grave confusione di idee con cui vi accostate al compito difficile e delicato di riformare il nostro diritto del lavoro. Il vero guaio è che non vi limitate a non affrontare i veri nodi cruciali della riforma necessaria, ma intervenite in modo episodico, disorganico, (il sottosegretario Viespoli lo ha riconosciuto). Non c'è un disegno riformatore chiaro che non sia quello di erodere sistematicamente le protezioni nell'area nell'area del lavoro debole, del lavoro di serie B o di serie C, accentuando il dualismo del nostro sistema, il regime di vero e proprio *apartheid* che separa i lavoratori protetti dai poco o per nulla protetti. Basta leggere il titolo caotico che è stato dato a questo disegno di legge per avere un'idea della sua disorganicità; quella disorganicità che, con notevole senso dell'umorismo, il relatore Maurizio Castro ha ribattezzato come «stratificazione normativa virtuosa»! Nell'autunno scorso, quasi contemporaneamente, l'11 e il 12 novembre, sono state rivolte al Governo due sollecitazioni per un ripensamento profondo del modo in cui si è fin qui legiferato, soprattutto ma ma non soltanto nella materia del lavoro: una dall'Unione europea e una dall'opposizione. L'Unione europea con il *Decalogue for Smart Regulation*, emanato a Stoccolma, ha invitato tutti i legislatori nazionali alla sobrietà e semplicità nella produzione delle norme legislative, alla cura della loro idoneità ad essere lette e capite da tutti i loro destinatari. L'opposizione, dal canto suo, ha presentato proprio qui in Senato, per la prima volta da un progetto di nuovo codice del lavoro organico in 70 articoli, con abrogazione di centinaia di leggi che oggi compongono la disordinatissima disciplina di questa materia (mi riferisco ai disegni di legge nn. 1872 e 1873 del 2009). La maggioranza per un verso si è mostrata totalmente indifferente, impermeabile a questi due segnali; per altro verso è andata avanti a testa bassa con questo disegno di legge-minestrone, di difficilissima lettura anche per gli addetti ai lavori, che costituisce davvero un esempio di scuola della cattiva qualità della legislazione. Alcune cose, certo, si leggono e capiscono molto bene in questo minestrone. È chiaro a tutti, per esempio, il passo indietro che viene compiuto con il comma 1 dell'articolo 14 rispetto al principio della trasparenza totale che solo un anno fa avevate accettato di inserire nella riforma Brunetta delle amministrazioni pubbliche. Sia ben chiaro, sul comma 2, che si riferisce ai rapporti di lavoro, siamo pienamente d'accordo e abbiamo cooperato alla sua stesura, ma il comma 1 abroga tutta la parte residua della norma e questo costituisce un passo indietro, un regresso secco rispetto a quanto era previsto da quella legge. È altrettanto chiaro a tutti il modo regressivo in cui avete ritenuto di affrontare il problema della povertà dell'offerta educativa attuale del nostro sistema per i giovani quindicenni che non proseguono gli studi. Invece di adottare misure capaci di allinearci con i Paesi più progrediti d'Europa, avete compiuto la scelta rinunciataria di abbassare di nuovo l'età dell'obbligo scolastico, facendo retrocedere ulteriormente il nostro Paese in una graduatoria europea nella quale già siamo in una posizione per nulla lusinghiera. È ancora chiaro a tutti l'enorme spazio che si apre a ogni genere di malversazione con la previsione della possibilità di compromettere in arbitri le controversie in materia di pubblico impiego al punto che nel momento stesso in cui questa norma viene varata, il Governo è costretto ad accogliere un ordine del giorno che lo impegna a emanare disposizioni per limitarne drasticamente l'applicazione.

parte degli arbitri, equivale a eliminare questa inderogabilità. Basta scegliere l'arbitro disposto a disapplicare la legge. Vorrei precisare a tal riguardo, collega Castro, che non è vero che l'arbitrato può essere attivato soltanto con il contratto certificato, come lei ci ha detto in quest'Aula. La legge che state approvando prevede l'attivabilità dell'arbitrato in qualsiasi momento della controversia. Non è vero che il certificatore ha la responsabilità di un controllo di merito sulla clausola compromissoria. Il certificatore ha la sola funzione di certificare la volontà negoziale delle parti e, se queste esprimono una volontà conforme a quanto previsto in questa legge, il certificatore non può negare la certificazione. Dunque, che cosa ci viene a dire il relatore a questo proposito? C'era una cosa importante che andava fatta in materia di arbitrato e che abbiamo invano proposto e riproposto in sede di emendamento: consentire che i contratti collettivi disponessero la soluzione arbitrale delle controversie relative a diritti nascenti esclusivamente dai contratti collettivi stessi. Questo sì che avrebbe segnato una svolta virtuosa, dimezzando il contenzioso giudiziale. Tutte le vertenze in materia di retribuzione o di inquadramento professionale avrebbero potuto essere oggetto della clausola collettiva compromissoria. Oggi, in Italia, il 47 per cento delle controversie riguarda proprio questioni retributive, a cui se ne aggiunge un 18 per cento in materia di inquadramento. Quindi, più della metà delle controversie giudiziali avrebbe potuto essere eliminata e passata alla competenza arbitrale. Ma, incomprensibilmente, avete rifiutato questa che sarebbe stata la vera riforma da fare per promuovere l'arbitrato nel nostro Paese. La cosa curiosa è che questa scelta è incomprensibile anche per voi, dal momento che non avete saputo indicare alcun motivo per il vostro rifiuto, e avete invece deciso di consentire la clausola compromissoria pattuita al livello individuale, della quale già detto. Norme come questa che state varando non verranno utilizzate dagli imprenditori seri, i quali non cercano scappatoie per aggirare i diritti dei loro dipendenti. Norme come questa allargheranno ancora un poco gli spazi marginali di elusione del diritto del lavoro. E questi spazi consentiranno di lucrare qualche rendita a qualche faccendiere in più. Ripeto che con ciò non mi riferisco né agli enti bilaterali nè alle organizzazioni sindacali, ma a chi organizzerà l'elusione al margine, con gli imprenditori meno seri. Non sono certo queste le riforme di cui il nostro sistema di relazioni industriali Ma quello che colpisce, in questo vostro modo di affrontare i mali che affliggono il nostro diritto del lavoro, sono gli esiti paradossalmente opposti a ciò che voi stessi vi proponete di conseguire, prodotti prodotti da quello che il senatore Castro magnifica come il metodo della "stratificazione normativa virtuosa". Due soli esempi. Incapaci di affrontare seriamente, organicamente, il problema dell'equilibrio tra libertà di impresa e responsabilità sociale dell'impresa, vi siete proposti un intervento furbesco di depotenziamento surrettizio del controllo giudiziale sulle scelte imprenditoriali in materia di giustificato motivo di trasferimento, licenziamento, organizzazione aziendale

avete compiuto questo intervento in modo così maldestro che, nel comma 3 dello stesso articolo 30, siete riusciti a infilare una disposizione che estende oltre ogni limite la discrezionalità del giudice, consentendogli di ergersi a unico interprete nientemeno che dell'«interesse oggettivo dell'organizzazione aziendale». In questo modo avete definitivamente espropriato non solo le imprese, ma anche il sistema stesso delle relazioni industriali, di ogni autonomia, attribuendo ai giudici lavoro un ruolo che non è attribuito loro su questo terreno in nessun altro Paese occidentale. Voi lo sapete bene, perché non solo le organizzazioni sindacali, ma anche Confindustria ed altre associazioni imprenditoriali hanno protestato per questo e hanno rilevato

Ancora peggiore è il pasticcio che avete fatto a proposito dell'articolo 32 sui contratti a termine, dove volevate sostituire la sanzione della reintegrazione e della conversione del contratto a tempo indeterminato ed invece avete aggiunto la sanzione indennitaria quella precedente. *( Brusìo).* Colleghi della maggioranza, credetemi, questi 50 articoli che state aggiungendo alle 2.000 pagine del nostro vetusto codice del lavoro non fanno fare al nostro tessuto produttivo alcun passo avanti. Ciò di cui abbiamo bisogno per rendere più organico, credibile e realmente applicabile universalmente il nostro diritto del lavoro per le nuove generazioni, per i nostri figli, che oggi il diritto del lavoro non lo vedono neppure da lontano, non è questo In attesa che apriate gli occhi noi, ovviamente, non possiamo che votare contro questo ultimo brutto capitolo della stagione delle mancate riforme del nostro mercato del lavoro.

senatore Giuliano. all'interno delle Commissioni che in Aula. Sono stati trattati temi molto delicati e sono sorte anche polemiche talvolta su presupposti di fatto non veritieri o, addirittura, quando ci si è accaniti in modo particolare sull'arbitrato evocando il problema dell'equità e paragonandolo ad una sorta di arbitrarietà. Evidentemente i due concetti sono assolutamente confliggenti e contrastanti, tanto è vero che in materia di equità sia il senatore Treu che il senatore Ichino sanno benissimo che ci si uniforma alle norme generali del diritto.

La 10ª Commissione permanente è dunque autorizzata a convocarsi domani, in sede deliberante, per la discussione del disegno di legge sul *Made in Italy*, già concluso